il seguito della discussione del disegno di legge n. 2541, già approvato dalla Camera dei deputati

Oggi, signor Presidente, legislature, approda al voto finale in questa Assemblea il disegno di legge di iniziativa parlamentare sui piccoli Comuni. È certamente un provvedimento che rappresenta un segnale di novità per le politiche del territorio

rappresentano una realtà importantissima per la difesa dell'ambiente, dell'agricoltura e dei beni culturali. Basti pensare che in essi si trova il 16 per cento dei musei, dei monumenti e delle aree archeologiche e vi si produce la gran parte dei nostri prodotti a denominazione d'origine riconosciuta. L'identità del Paese è costituita dai mille campanili; una realtà messa però in discussione dal fenomeno dello spopolamento, che non conosce sosta e mette a rischio la stessa sopravvivenza dell'eccezionale diversità culturale, vera ricchezza Aveva ben intuito il rischio esiziale insito nei fenomeni di abbandono del territorio il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, tragicamente assassinato nell'esercizio delle funzioni a causa delle sue battaglie ambientaliste e di difesa del territorio. Fermare l'emorragia di giovani, invertire la tendenza all'abbandono dei centri storici minori, ridare vitalità e produzione ai terreni agricoli abbandonati, fornire incentivi per il rilancio turistico dei piccoli borghi (che sarebbe per noi una ricchezza immensa), valorizzare gli itinerari storici e quelli religiosi, che passano per le aree interne; sono queste alcune delle scommesse che potrebbero realmente cambiare il modello di sviluppo del Paese. L'importante è capire in che direzione deve andare l'Italia. Se si vogliono valorizzare gli itinerari nell'Italia minore e lo sviluppo sostenibile dei piccoli centri abitati, o proseguire sulla strada del consumo di suolo e di quelle «grandi opere» che hanno generato, troppo spesso, cattedrali nel deserto. Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare affronta alcune delle problematiche di fondo che caratterizzano le difficoltà di sopravvivenza dei piccoli Comuni.

Purtroppo, non con moltissime risorse. Di rilievo anche le disposizioni per favorire la diffusione della banda larga per aiutare a togliere dall'isolamento i piccoli Comuni, su cui nessuno investe perché non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce, il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore del servizio postale per promuovere la riapertura di tutti gli uffici postali dismessi, le iniziative per promuovere il consumo e il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari cosiddetti a chilometro utile e certamente questa è una nuova ed interessante definizione che ritengo potrà trovare in futuro applicazione anche in provvedimenti di altra natura. Sono certamente apprezzabili, anche se meritavano ben altro impegno finanziario, le misure per il recupero dei centri storici e per contrastare l'abbandono dei terreni, mentre rappresentano un tentativo lodevole di invertire una tendenza purtroppo radicata le disposizioni volte a favorire la diffusione della stampa quotidiana e a promuovere la realizzazione di produzioni culturali e cinematografiche anche nei piccoli Comuni. Nel complesso, quindi, si tratta di un provvedimento di buon senso, il cui contenuto è stato certo arricchito e migliorato nel corso della lunga gestazione parlamentare, ma che rappresenta, a nostro giudizio, solo un barlume di novità in un quadro complessivo delle politiche territoriali che va in tutt'altra direzione. il binario morto nel quale l'Esecutivo e la maggioranza hanno deliberatamente instradato il disegno di legge sul consumo di suolo, tuttora all'esame del Senato, e l'assenza di impegni finanziari adeguati, anche nelle prospettive delineate dal DEF, per il risanamento idrogeologico del Paese e per il contrasto ai cambiamenti climatici. Voglio ricordare anche la necessità di mettere in sicurezza il nostro patrimonio edilizio, a cominciare da quello più prezioso dei centri storici, nei confronti del rischio sismico, e le conseguenze drammatiche che il mancato adeguamento produce nel caso di eventi calamitosi, incrementando la tendenza preoccupante allo spopolamento delle aree interne. In direzione opposta a quanto sarebbe necessario è indirizzata anche la politica energetica del Governo, di fatto rivolta a rallentare la crescita delle energie rinnovabili che potrebbe invece trovare proprio nei piccoli Comuni una prospettiva di sviluppo di assoluto rilievo, così come deludente e, per certi aspetti, controproducente, è il disegno di legge sulle aree naturali protette, attualmente in discussione in Commissione ambiente. Pertanto, non sono certamente sufficienti i 15 milioni di euro all'anno, stanziati da questo disegno di legge, per il Fondo strutturale dedicato ai piccoli Comuni per invertire un quadro complessivo di politica territoriale che non ci convince affatto e che porta con sé le stimmate dell'arretratezza, non certo quelle del nuovo modello di sviluppo che pur sarebbe necessario e urgente promuovere, anche sul fronte dell'occupazione.

Signor Presidente, l'*iter* di questa proposta di legge è iniziato nel 2014 e da allora, soprattutto alla Camera, è stato condotto da parte del Movimento 5 Stelle un lavoro incessante di ascolto e confronto, con incontri dei rappresentanti delle diverse e variegate realtà che hanno a cuore il destino delle piccole comunità. Non è un caso infatti che dopo quattro legislature in cui questa legge è stata arenata, si sia riusciti oggi, con l'apporto decisivo del Movimento 5 Stelle, a farla approvare e speriamo naturalmente Ma partiamo dal contesto. Quando parliamo di piccoli Comuni, ci riferiamo al 70 per cento dei Comuni italiani, che ha una popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti. Questi Comuni occupano il 54,4 per cento del territorio italiano e in essi risiede il 16,6 per cento della popolazione totale. Si tratta di oltre 10 milioni di persone. Per capire se il disegno di legge si muove nella direzione giusta, dovremmo quindi chiederci: quali sono le esigenze di queste amministrazioni locali? Sicuramente i piccoli paesi non hanno bisogno di grandi opere infrastrutturali di superappalti; essi hanno invece bisogno di riattivare la piccola e media impresa, partendo dagli artigiani e dagli agricoltori. Hanno bisogno di ripartire dalle piccole cose, c'è la necessità che si ponga l'attenzione sulle persone e sui loro effettivi bisogni. Negli ultimi quattro anni, sulla base della legislazione sul contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica (la cosiddetta *spending review*), è stato operato un drastico taglio lineare sul sistema dei servizi urbani legati alla gestione amministrativa del territorio. Parliamo dei servizi minimi, dal settore sanitario al settore scolastico, ai servizi postali e di trasporto. È del tutto conseguente che questa drastica diminuzione dei servizi abbia comportato un sempre più preoccupante crollo delle attività economiche private. Passeggiando per un piccolo Comune purtroppo si leggono soltanto avvisi di vendita e chiusura di attività. Il testo unificato, già approvato alla Camera dei deputati esattamente un anno fa, il 28 settembre 2016, vuole fornire una risposta all'abbandono; esso tenta di fornire strumenti per avviare questa imponente opera di ricostruzione. È un testo unificato condiviso da tutti. Sicuramente si poteva fare di più, se solo il Governo avesse voluto. Considerato che, come detto, stiamo parlando di una realtà che coinvolge il 54,4 per cento del territorio italiano, è evidente che, prevedendo misure che ne favoriscono la ricostruzione, tutto il Paese ne trarrà beneficio. Con riferimento all'articolato, di particolare rilievo sono gli articoli 4 e 5, che prevedono le misure necessarie al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, con attenzione in particolare al tema del consolidamento statico e antisismico degli edifici, tema purtroppo tristemente attuale. Il recupero dei piccoli borghi potrebbe rappresentare in questo modo anche un'imperdibile opportunità per mettere in sicurezza la parte più fragile del nostro patrimonio immobiliare. I piccoli borghi sono molto spesso la culla di prodotti tradizionali, sede di prodotti enogastronomici con marchi di qualità. Sono quindi questi gli ambiti sui quali far leva per il rilancio delle attività produttive di questi luoghi e proprio su questi aspetti si basano i contenuti degli articoli 10 e 11; articoli da noi fortemente voluti ed infine ottenuti, articoli che riguardano non solo la promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile, ma anche misure atte a favorire la vendita diretta di tali prodotti, come ad esempio prevedere all'interno delle strutture commerciali degli spazi dedicati appunto ai prodotti del territorio. Quindi, attenzione alla comunità, al patrimonio immobiliare e alle attività produttive. Tutto questo però non basta, se i piccoli borghi restano privi dei servizi essenziali che consentono di godere appieno dei ritmi che solo in questi luoghi si possono sperimentare. Gli articoli 8, 9 e 13 cercano proprio di colmare queste carenze. Parliamo di servizi essenziali quali la scuola, i trasporti e la possibilità di effettuare pagamenti di imposte, tasse e tributi. Siamo riusciti ad inserire in questo provvedimento, all'articolo 3, anche lo sviluppo dei cammini storici, un importante volano per il rafforzamento e lo sviluppo del turismo di questi luoghi ricchi di storia e cultura. Il tutto con un finanziamento di 3 milioni di euro. L'entità degli stanziamenti previsti nel provvedimento poteva essere senz'altro maggiore, con un po' più di coraggio soprattutto da parte del Governo. Avrebbero potuto essere inserite altre proposte che erano state avanzate dal Movimento 5 Stelle e non solo. Il testo presenta ancora delle lacune: ad esempio, non ci sono misure volte a favorire i servizi sanitari destinati alle aree rurali e montane, né sulla gestione delle risorse idriche o sulla diffusione delle fonti di energia rinnovabile e dell'efficientamento energetico. Qui in Senato le proposte del Movimento 5 Stelle avevano l'obiettivo di calibrare e colmare queste lacune ma, seppure con valutazione non ostativa da parte della Commissione bilancio, non sono state accolte, anche per evitare che il provvedimento, per l'ennesima volta, si arenasse e non venisse approvato. Penso ad esempio all'emendamento 12.0.2, che, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, prevedeva l'avvio in via sperimentale proprio nei piccoli Comuni, anche in forma associata, del sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale, servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici. Si tratta di una semplice proposta, che però potrebbe essere molto importante nei piccoli centri, perché andrebbe a ridurre in maniera considerevole la percentuale dei rifiuti prodotta. Tuttavia questa nostra proposta è stata accolta dal Governo con l'approvazione di un ordine del giorno che prevede, fra l'altro, l'impegno ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, per l'attivazione di misure per la riduzione degli imballaggi, anche attraverso progetti sperimentali per ridurre l'utilizzo di contenitori e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili dalle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici, così come fra l'altro abbiamo proposto in un disegno di legge a mia prima firma, l'Atto Senato 2804, che purtroppo temo giacerà in un cassetto fino alla fine della legislatura. Come già detto, il testo non è perfetto e di certo poteva essere migliorato, ma rappresenta comunque un piccolo, ma importante passo verso la ricostruzione dei piccioli Comuni e non volendo rischiare di vederlo nuovamente rinchiuso in un cassetto, il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà voto favorevole Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame avvia un percorso per valorizzare e riconoscere il ruolo importante che rivestono i piccoli Comuni per la comunità italiana. Riteniamo infatti che il disegno di legge, a cui andrà il voto favorevole del nostro Gruppo, rappresenti solo un primo, timido passo nella valorizzazione del ruolo dei piccoli Comuni nel contesto nazionale, cui dovranno seguire ulteriori disposizioni che ne salvaguardino la peculiarità e garantiscano un contesto normativo, che semplifichi gli adempimenti e garantisca un adeguato livello di finanziamenti. Si stanziano complessivamente 100 milioni di euro in sette anni:

Troppo spesso sentiamo accostati al piccolo Comune concetti come "fuga dal territorio", "periferia del Paese", "problemi di bilancio" e potrei continuare. Il piccolo Comune non è un problema e non è un ente inutile: rappresenta invece una risposta a problematiche di interesse generale, legate al dissesto idrogeologico, all'offerta turistica, alla tutela paesaggistica culturale e via dicendo e anche alla richiesta di elevati *standard* di qualità della vita. II provvedimento in esame è un contenitore atto ad evidenziare numerosi principi condivisibili, ma il ragionamento deve essere completo e molto più articolato. Ogni contenitore che si rispetti per definizione deve essere riempito, altrimenti con il passare del tempo prenderà le sembianze di semplice scatola vuota.

Proprio per questo motivo abbiamo proposto in fase emendativa almeno il raddoppio degli stanziamenti. Le problematiche maggiori di ogni ente locale sono di far fronte ad una molteplicità di azioni e di funzioni, con risorse economiche sempre più limitate. Quindi, le risorse aggiuntive di cui stiamo parlando non sono in grado di cambiare radicalmente le condizioni di tali soggetti. Il mantenimento dei servizi, il riconoscimento delle difficoltà, la valorizzazione delle peculiarità di questi piccoli enti richiedono risorse certe per intraprendere una corretta e strutturata politica di governo del territorio. Non possiamo negare che ci saremmo aspettati qualcosa in più. Gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo in Commissione e in Assemblea erano volti proprio a rendere il provvedimento più aderente alla realtà attuale. qualche ulteriore esempio, in aggiunta a quanto evidenziato dai senatori Ceroni e Malan in discussione generale. Al comma 2 dell'articolo 1, leggendo i diversi requisiti richiesti ai piccoli Comuni per beneficiare dei finanziamenti

«significativo decremento della popolazione» o «disagio insediativo» o «inadeguatezza dei servizi essenziali»? Non crediamo possibile che il Parlamento si esima, come ha fatto in questa occasione, dal fornire dettagliate informazioni al Governo con indirizzi chiari e non aleatori. Guardando, poi, ai contenuti del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni,

Una diversa impostazione avrebbe consentito di evitare i relativi oneri amministrativi e operativi. Ancora, ad esempio, sarebbe stato opportuno inserire la previsione secondo cui nel Piano nazionale venisse garantita ai piccoli Comuni, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni in generale, idroelettriche in particolare, una riserva di acquisizione delle stesse nonché una previsione atta a favorire l'acquisizione di quote di proprietà di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da far sì che i piccoli Comuni potessero introitare risorse e avere finanziamenti su questo versante. Non abbiamo visto nulla di ciò. Non vediamo nemmeno una semplificazione in merito a pesanti adempimenti di bilancio cui sono sottoposti i piccoli Comuni italiani, quantomeno prevedendo che gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non siano tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione, pesantissimo adempimento: strumento inutile per programmare, dato che la cosiddetta programmazione nei piccoli Comuni si è sostanzialmente ridotta al nulla. All'articolo 2, ancora, non si comprende cosa c'entri l'ente parco per promuovere nei piccoli Comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, confusionaria sovrapposizione di ruoli che francamente ci fa dubitare dell'esperienza amministrativa di chi ha scritto questo passo della norma. Inoltre, come è possibile che tra gli obiettivi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, istituito all'articolo 3, non sia esplicitamente inserito l'obiettivo - priorità delle priorità - del contrasto allo spopolamento? Lo spopolamento è un'autentica piaga che affligge la gran parte dei piccoli Comuni, perlopiù di natura montana, con percentuali di riduzione della popolazione, negli ultimi anni anche superiori al 30 per cento, e contestuale migrazione - lo sappiamo - dei giovani verso altre terre. La vera scommessa dovrà essere quella di prevedere norme che sostengano un controesodo verso i piccoli Comuni. È necessario attivare disposizioni che prevedano incentivi di tipo fiscale con agevolazioni sulle addizionali Irpef comunali e sulle imposte sulla casa, per favorire il ritorno di residenza verso i territori di cui stiamo parlando. Da qui anche la necessità di affrontare nel provvedimento il tema delle differenze esistenti tra piccoli Comuni di pianura e piccoli Comuni di montagna, attraverso un'intelligente politica amministrativa, economica e finanziaria incentrata sul riequilibrio, ove necessario. Oggi, signor Presidente, si parla di questo provvedimento come necessario per la sopravvivenza dei piccoli Comuni, ma noi non vogliamo vedere i piccoli Comuni sopravvivere; li vogliamo vedere vivere pienamente, nell'effettiva possibilità di esprimere programmazione e gestione corrispondenti pienamente, appunto, alle richieste di sviluppo di territorio, cittadini e famiglie. Se intendiamo questo provvedimento come l'inizio di una partita più grande e importante da giocare, allora ci siamo, e dovranno necessariamente seguire interventi sin dalla prossima legge di bilancio sulla *governance*, sui servizi, sulle risorse, nel segno del realismo e della concretezza. Se, però, con questa approvazione ci illudiamo di aver fornito risposte risolutive all'articolata problematica, la realtà ben presto ci metterà nuovamente di fronte a ulteriori peggioramenti della situazione generale e dei concreti e quotidiani problemi che affliggono i piccoli Comuni italiani, tanto più che l'impossibilità di emendare il testo - cui ci ha costretti la maggioranza ci consegna un provvedimento poco accurato e addirittura, a tratti, frettoloso. Voteremo favorevolmente, consapevoli che la materia dovrà essere oggetto di ulteriore impegno, dato che l'attuale approccio lascia irrisolte molte questioni di non secondaria importanza per la vita di chi abita e opera nei piccoli Comuni, risorsa e non problema per il nostro Paese.

dopo l'approvazione della legge sugli ecoreati e di quella sulla agenzie ambientali, per la terza volta in questa legislatura ci apprestiamo a votare un disegno di legge di iniziativa parlamentare che avrà ricadute importanti su ambiente, economia e cultura. un provvedimento necessario, di cui si discute da tempo (da ben tre legislature), frutto dell'ascolto e del dialogo tra i diversi Gruppi parlamentari e dell'ottimo lavoro fatto dai colleghi della Camera dei deputati - a partire da Ermete Realacci, che ne è stato da sempre sostenitore - che hanno concorso alla stesura di un testo condiviso, votato da un'ampia maggioranza. A onor del vero, signor Presidente, credo sia importante sottolineare anche un altro aspetto. Se

Come ricordavo poc'anzi, con l'approvazione del provvedimento in esame inseriamo un altro tassello a quel quadro complessivo di riforma con cui, in questa legislatura, stiamo cercando di fornire nuove e più efficaci risposte ai temi della tutela dell'ambiente e della salvaguardia e valorizzazione dei territori, soprattutto dell'entroterra. L'intento che ci siamo prefissi - lo abbiamo detto più volte è il superamento dell'approccio alla sola risposta all'emergenza, passando a quello della pianificazione e programmazione di politiche di prevenzione nella gestione del territorio. il susseguirsi, con sempre maggior frequenza, di eventi calamitosi ci mette alle strette rispetto all'indifferibilità di fare della prevenzione il principale *asset* strategico su cui il Paese deve puntare nei prossimi anni. questi argomenti si rischia sempre di cadere vittima della retorica, ma vi assicuro che non è questo il caso. La comunità politica è ben consapevole della fragilità del nostro territorio sotto il profilo geologico, a cui si sommano l'incuria, l'abbandono, l'abusivismo e il consumo grazie a questa nuova consapevolezza, che ha sconfitto - questo sì - vecchi scetticismi, in quest'Assemblea siamo riusciti insieme a raggiungere importanti risultati, che hanno posto l'attenzione su temi centrali per nuovi modelli di sviluppo che possono creare valore e futuro. Si è già detto e scritto molto, ma desidero sottolineare che con il provvedimento in esame miriamo ad agire su una delle principali cause del dissesto idrogeologico, ossia lo spopolamento delle aree, soprattutto interne, e la relativa incuria dei territori. L'insediamento e il reinsediamento all'interno di questi luoghi è una risorsa per l'intera collettività nazionale, perché presidiare queste zone significa svolgere una funzione nell'interesse - sì - delle realtà circoscritte, ma anche di quelle che non appartengono a quel bacino a quella peculiare area geografica, ma al Paese intero. Attenzione, allora, a non cadere nella trappola del provvedimento campanilistico, fatto solo per pochi Comuni e che parrebbe avere, come ci è stato detto in passato, anche l'ambizione di un riordino istituzionale. Vorrei sottolineare che i piccoli Comuni sono un segmento molto rilevante del nostro Paese: i Comuni con meno di 5.000 abitanti sono 5.627 (pari coprono 160.000 chilometri quadrati (cioè il 54 per cento della superficie del nostro territorio) e ospitano poco più di 10 milioni di abitanti (cioè poco meno del 17 per cento della popolazione totale). Vi è poi il tema del recupero, della valorizzazione e della riqualificazione dei nostri tema drammaticamente portato all'attenzione dagli eventi del terremoto. Il lavoro che, come Parlamento e Governo, stiamo facendo va in questa direzione, Signor Presidente: da "Casa Italia" alle norme contenute nel collegato ambientale, alla proroga dell'ecobonus, esteso anche alle dotazioni antisismiche per case e condomini, ma soprattutto alla legge del consumo del suolo. Volevo dare una notizia al Senato: la prossima settimana sarà depositato il testo unificato unificato e cominceremo la procedura. Mi auguro che il testo possa essere approvato prima della fine della legislatura. Qualcuno ha detto che, per essere un provvedimento così ambizioso, è leggero dal punto di vista finanziario: si parla di 100 milioni di euro in più anni, destinati soprattutto alle comunità che sono in maggiore difficoltà. Ma, vedete, per sgombrare il campo da ulteriori polemiche, con questa norma stiamo definendo un'idea di Paese. E nel definire su cosa vogliamo investire nel prossimo futuro, apriamo un apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato, un capitolo che potrà essere rimpinguato a partire già dalla prossima legge di stabilità. Lavoriamo tutti assieme per poter rimpinguare questo capitolo. L'idea di Paese sul quale vogliamo puntare è quella rappresentata da questi borghi, elementi fondamentali - come avete detto in molti - della nostra identità, caratterizzati da un'elevata qualità della vita e da una forte coesione sociale, che racchiudono una parte molto importante del nostro patrimonio storico, artistico e paesaggistico e custodiscono molte molte eccellenze del sistema produttivo italiano. Nel corso di questi anni abbiamo visto moltiplicarsi con successo, ad esempio, delle forme di turismo dolce, cammini storici, percorsi ciclistici; abbiamo inoltre visto crescere una imprenditoria giovane, soprattutto in agricoltura, che scommette sulla qualità e sull'identità del territorio. Vorrei ricordare che il 93 per cento delle DOP e delle IGP ha a che vedere con i piccoli Comuni e il 79 per cento dei vini di maggiore qualità proviene dai territori dei piccoli Comuni. Dobbiamo sostenere queste potenzialità, superando gli squilibri: questa è la missione della legge. Vedete, cari colleghi, prima di fare il parlamentare, sono stato un presidente di parco e un sindaco e ho potuto toccare con mano i punti di forza e quelli di debolezza del nostro Paese. Volevo anche rassicurare gli amici di Forza Italia e i colleghi della Lega Nord, i quali dicono che i disastri sono successi solo adesso:

del Partito Democratico: è importante dirlo per onorare la verità. Con questo disegno di legge si cerca di accorciare le distanza tra i territori italiani e si affronta uno sforzo comune per costruire le condizioni e le opportunità, affinché questa parte dell'Italia possa realmente scommettere su di sé; affinché le nuove aziende che si svilupperanno possano competere nel mondo, grazie alla banda larga, alla qualità dei loro prodotti, al sincero entusiasmo di chi ci lavora e lì ha voglia di costruirsi un percorso di vita. Incentivare l'incontro tra tradizione e futuro e portare le comunità locali a fare più sistema, a intraprendere quei percorsi innovativi, ma anche più remunerativi, come la *green economy*, il turismo sostenibile o, ancora, puntando sull'agroalimentare di qualità e la filiera corta, fatta di buone pratiche, trasparenza e legalità. Tra le priorità - è bene ricordarlo - il provvedimento individua l'obiettivo di favorire la residenza nei piccoli Comuni, sia dei cittadini che delle attività produttive, partendo dal principio che l'insediamento è considerato una risorsa a presidio del territorio. In questo senso,

In particolare, su scuole e trasporti i piani nazionali dovranno tenere conto delle esigenze dei piccoli Comuni e delle aree rurali e montane.

le classi per i propri figli. E se proprio c'è da razionalizzare e da chiudere qualche classe, lo si faccia nelle città. Si prevede la possibilità di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio dal punto di vista della della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie originarie. È importante recuperare, conservare e rendere appetibili i centri storici. Si compie

sono poi azioni di sistema che mirano alla co-pianificazione, alla solidarietà e alla sussidiarietà. che dialoga e si completa con quella sulle aree protette, che mi auguro possa essere approvata definitivamente nelle prossime settimane e sui il Senato sta lavorando da qualche anno. Penso che l'Italia che vuole scrollarsi di dosso questo sentimento di indolenza che, spesso e ingiustamente, gli viene attribuito, può trovare in questo testo - se verrà approvato ed io me lo auguro - uno strumento utile per cercare nelle sue radici le energie per rinforzare le proprie ali. Sono queste,

Colleghi, chi vuole allontanarsi dall'Aula, è pregato di farlo in tempi rapidi.

nostro Paese. Mi riferisco al fatto che l'Agenzia europea del farmaco (EMA), un organo decentrato dell'Unione europea con sede a Londra e circa 1.000 dipendenti, che ha come compito principale quello di tutelare e promuovere la sanità pubblica, la tutela degli animali, mediante valutazione e controllo dei medicinali per uso umano, possa trovare sede in Italia. L'EMA è responsabile, in via principale, della valutazione scientifica delle domande finalizzate ad ottenere l'autorizzazione europea di immissione in commercio per i medicinali.

in un altro Paese dell'Unione europea. La riflessione che vogliamo fare oggi, e che credo sia davvero importante, è che l'Italia, che rappresenta uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea ed è uno dei più importanti Paesi produttori di farmaci, possa diventare sede di questa agenzia. In particolare, il riferimento è alla Lombardia, prima Regione italiana nel settore della produzione del farmaco con 28.000 addetti, più altri 18.000 persone che lavorano nell'indotto e dove ogni anno si investono sette miliardi di euro in ricerca e innovazione. Ecco, quindi, la grande possibilità di esercitare anche oggi, con il nostro voto, una pressione affinché la candidatura del nostro Paese venga presa seriamente in considerazione. Poi vedremo i motivi su cui fondiamo questa richiesta. Devo fare un passo indietro, per dire che il Gruppo di Forza Italia ha chiesto fin dall'inizio che l'EMA fosse nelle priorità del Governo in seguito alla Brexit. Voglio qui ricordare velocemente due passaggi. nelle comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo, proprio la mozione di Forza Italia, avente come primo firmatario il senatore Paolo Romani, chiedeva al Governo di porre in essere tutte le iniziative utili affinché l'EMA potesse venire in Italia. Poi siamo voluti tornare su questo tema nelle comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno. Sempre con una mozione, chiedevamo che tutto quanto poteva essere nelle disponibilità del Governo fosse fatto affinché la candidatura italiana avesse quel peso importante che vi ho illustrato qualche minuto fa. fa. Personalmente, io ho portato avanti fin dall'inizio questa iniziativa. In particolare, il 2 febbraio ho presentato la mozione,

pressione del presidente del Parlamento europeo Tajani che il 31 agosto, incontrando Guido Rasi, il direttore esecutivo dell'EMA (un italiano in un posto di eccellenza) ha evidenziato come fosse necessario che la selezione della nuova sede dell'agenzia avvenisse in a criteri oggettivi. garanzia che l'agenzia sia pienamente operativa nel momento in cui dovrà lasciare Londra e il Regno Unito. Per questo, il Presidente della Regione Lombardia, Maroni, ha messo subito a disposizione un palazzo della Regione, il palazzo Pirelli, proprio

Milano è in grado di offrire, anche con sedi eccellenti come quella di Varese, collegata all'ISPRA, agli studenti la possibilità di un percorso formativo europeo,

del Parlamento italiano in sede europea per dire che Milano ha i requisiti; vuole EMA; vuole questa importante Agenzia e questa importante opportunità di sviluppo per il nostro Paese.

questo *input* al Governo. Ovviamente dal 2 febbraio il tempo è passato e, pertanto, penso sia opportuno variare leggermente il dispositivo e dire di proseguire il percorso di sostegno alla candidatura perché il Governo ha già costituito il *dossier* che ottempera ai sei requisiti individuati

hanno una caratteristica unica che non tutti i ricercatori hanno: la capacità di risolvere i problemi quando vengono posti nella ricerca. I ricercatori italiani sono preferiti dalle aziende del farmaco nel mondo per la loro capacità di essere rigorosi

problemi. Per questo motivo penso sia importante riproporre il modello Expo: un gioco di squadra che dia all'Italia la possibilità di offrire tanti posti di lavoro nel nostro Paese - e ne abbiamo davvero bisogno - un'opportunità ulteriore di crescita per ridire che l'Italia in Europa ha un posto centrale

avanzata dall'Italia per avere nel Paese e, segnatamente, a Milano la sede dell'Agenzia europea del farmaco sia un impegno che coinvolge l'intero Parlamento. Non vi è dubbio che il Governo abbia già iniziato da tempo un'azione importante di promozione della candidatura

è importante però che si agisca anche con una diplomazia parlamentare. Da questo punto di vista, la formazione di un intergruppo parlamentare italiano ed europeo in grado di promuovere nelle sedi parlamentari la candidatura dell'Italia è un fatto rilevante, che vorrei noi cogliessimo in tutta la sua portata. Il terzo elemento, anch'esso una novità, è il fatto che sta agendo anche e finalmente una diplomazia dell'impresa e delle aziende per favorire il successo della candidatura dell'Italia e di Milano per

lo sviluppo di un Paese avviene a rete; vi è dunque un coinvolgimento dell'intero Paese, la promozione e l'avanzamento dell'impresa farmaceutica riguarda l'intero Paese, anche se Milano e la Lombardia hanno uno dei più importanti

Technopole, che mi auguro comincerà a marciare tra poco tempo e sarebbe il primo centro europeo di lavoro e ricerca sulla genomica e sui *big data*.

dico che avere EMA a Milano significherebbe

la farmacosorveglianza, sia uno dei punti più importanti per la sicurezza dei cittadini rispetto ai farmaci che vengono assunti. La produzione di farmaci richiede anche una sperimentazione adeguata e appropriata. appropriata. La relazione con le imprese sul piano dei prezzi è l'altro grande tema che appartiene ad EMA. Non nascondo, come abbiamo detto in tante occasioni, che abbiamo anche bisogno di segnalare che il farmaco non è una merce come le altre, che i prezzi (particolarmente dei farmaci innovativi) crescono anno dopo anno e che noi abbiamo bisogno di un un soggetto unico europeo in grado di trattare con i colossi del farmaco. Avere EMA a Milano significa per noi avere un'opportunità in più.

di accogliere una residenza pregiata come quella dei ricercatori e dei funzionari di EMA. Penso a una sede di straordinario prestigio come è il grattacielo Pirelli, una delle opere più straordinarie, che non a caso è stata anche sede della Regione, a segnalare che Regione e Comune si associano e promuovono, assieme alle istituzioni nazionali, la candidatura di Milano come sede dell'EMA. Molto importante, l'abbiamo fatto per Expo: ognuno può pensare quel che vuole, forse è stato giusto, forse è stato sbagliato, ma io credo sia stata una scelta vincente. Ci sono momenti in cui il Paese

modernità con l'umanità, e questo è un punto non irrilevante, che mi rende orgogliosa di essere milanese e che deve rendere orgogliosa l'intera Italia. Si potrebbe ancora parlare a lungo, ma credo che per noi parleranno meglio i nostri colleghi che andranno in giro per l'Europa a interloquire con i Parlamenti; i Ministri e il presidente Gentiloni, che incessantemente stanno lavorando; il presidente Maroni e il sindaco Sala, a loro volta impegnatissimi insieme in questa

di Milano come sede dell'agenzia regolatoria europea del farmaco. Insomma, lo dico con uno *slogan* finale: dobbiamo batterci insieme e sperare. La competizione è molto aspra, dovete saperlo, e vogliamo la trasparenza dei risultati. Vogliamo che i risultati siano trasparenti perché non vorremmo mai che fossero altri i criteri rispetto all'appropriatezza per definire la nuova sede dell'Agenzia europea del farmaco. Dobbiamo batterci insieme per la trasparenza e perché il sistema perché il sistema Paese possa fare un passo in avanti. Insomma, se vince Milano, vince l'Italia e credo che questo punto debba renderci orgogliosi e uniti.

affinché l'obiettivo di portare a Milano la sede dell'agenzia europea del farmaco abbia successo. Ricordo peraltro che ad un precedente disegno ad un precedente disegno di legge avevamo affiancato un nostro ordine del giorno che impegnava il Governo in tale direzione, quindi questo è un percorso che vogliamo rimarcare in maniera forte, anche con una mozione

la Regione Lombardia, il Comune di Milano e, come abbiamo potuto vedere anche nei giorni scorsi, il Ministro della salute, quindi il Governo, affinché possa avere successo. Chiunque sostenga questo progetto per noi è soggetto politico gradito. Cosa si chiede? Che l'Italia faccia la propria parte presso la Commissione europea affinché, dopo la Brexit,

Stiamo parlando della realtà produttiva più importante del Paese, soprattutto legata al settore della ricerca farmaceutica. Ricordo peraltro che, come pubblicato anche da Assolombarda, nel 2015 sono stati pubblicati ben 11.600 articoli scientifici, dei quali 6.200 nel campo nel campo della scienza della vita, e questo solo a Milano. Si tratta quindi un *unicum*. Il contesto politico ovviamente dev'essere favorevole in tutta Europa: è chiaro che non si possono aspettare casualità e bisogna lavorare affinché queste opportunità si verifichino.

Non stiamo parlando quindi di qualcosa di secondario; credo infatti che quando si parla di posti di lavoro non si possa che trovare massima convergenza. Occorre però un'azione politica molto forte in sede europea. Francesi e tedeschi si mettono d'accordo molto facilmente. Il Governo deve entrare in maniera opportuna in questi equilibri e fare in modo che non per scelta politica, ma squisitamente per il merito, non esista sede europea migliore rispetto a quella proposta

dopo Londra, Milano sia la città più idonea in assoluto. Sono convinto che il presidente Gentiloni, non solo con Macron, ma anche con gli altri

in una riunione ufficiale nel settembre 2016, a seguito di un vertice tra il Presidente della Regione Lombardia, il sindaco di Milano ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali

sia una conquista dell'intero Parlamento italiano, ovviamente ben rappresentato in questo campo dal Governo.

anche se dobbiamo rimarcare, come ho detto ieri, l'inutilità di questo dibattito, visto che tutto il Paese è d'accordo (sindaco, Regione e Governo), che la candidatura è già stata messa in atto e che il Governo ha già stanziato 59 milioni di euro.

ci si attrezzi per costruire qualcos'altro. Ebbene, con questo ordine del giorno noi chiediamo che le amministrazioni competenti vengano impegnate a non costruire ulteriormente a Milano, che di cemento forse ne ha a sufficienza ed avrebbe bisogno di altro, di alberi Un altro aspetto importante che sottolineiamo nell'ordine del giorno è che la gestione di tutto ciò che ruota intorno a quest'Agenzia in futuro avvenga con trasparenza.

di connessione con il territorio e con le aziende che a quelle agenzie fanno riferimento che non sono sempre sani. Oggi si è parlato solo della bellezza di avere un'agenzia nel territorio, che è più di altri sviluppato nel settore farmaceutico e della biomedicalità, ma ci si dimentica di dire che forse questa Agenzia, nel momento in cui si innesta in questo territorio potrebbe subire

che nell'industria del farmaco vede il suo settore di punta. Pertanto le raccomandazioni che facciamo al Governo con questo ordine del giorno sono di vigilare sui meccanismi di trasparenza, sull'utilizzo dei fondi e sulla non costruzione di

Signor Presidente, colleghi, intervengo con molto piacere nella discussione per supportare la candidatura di Milano a ospitare l'Agenzia europea del farmaco, non solo perché ha le migliori caratteristiche e potenzialità per ospitare l'EMA, ma soprattutto perché credo che questa sia la scelta più strategica dal punto di vista economico e politico che l'Italia possa portare avanti in questi mesi in Europa. L'eventuale arrivo nel capoluogo lombardo dell'Agenzia europea del farmaco potrebbe portare un indotto di oltre un miliardo di euro (ben 890 persone lavorano nell'Agenzia), per non parlare poi dell'incremento qualitativo che la ricerca tecnologica italiana avrebbe qualora fosse completamente operativa l'intera struttura scientifica di supporto. Il mio auspicio, con un voto unanime dell'Assemblea, è che la candidatura di Milano sia più forte, come è più forte la convinzione che di fronte a noi abbiamo un'opportunità di sviluppo in termini di ricerca, medicina e innovazione. Sia il presidente del Consiglio Gentiloni Silveri che il presidente del Parlamento europeo Tajani hanno sottolineato che la candidatura, sebbene difficile e in salita, ha tutte le possibilità, nonché i criteri oggettivi, per essere favorita. Ecco perché mi auguro che anche il Parlamento faccia la sua parte, approvando magari un'unica e condivisa mozione, che vada oltre le capricciose e irragionevoli argomentazioni che nulla hanno a che fare con una sfida sul futuro dell'Italia. È importantissimo mostrare un Paese unito che supporta la candidatura di Milano. mi auguro che il voto di oggi sia appunto unanime e a favore di questa candidatura. Ci sono ben 19 candidature e i nostri concorrenti sfrutteranno ogni nostra possibile criticità. L'incertezza politica legata ai prossimi voti nazionale e regionale nel 2018 potrebbe essere strumentalmente usata contro la candidatura di Milano. Ecco perché è fondamentale mostrare l'unità e la compattezza di tutte le forze politiche in favore di Milano. La presentazione della candidatura lo scorso 25 settembre a Bruxelles è stata unitaria. Erano presenti il ministro Lorenzin, il sottosegretario Gozi, il presidente Maroni e il sindaco Sala: differenti ruoli e differenti parti politiche, ma unione e unità di intenti nel promuovere Milano quale futura sede dell'EMA. Rivolgo quindi un appello in particolare ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che in questo aspetto hanno un ruolo decisivo. Un loro voto contrario o anche solo di astensione o una loro incertezza verranno valutati molto negativamente e usati contro l'Italia da parte dei nostri concorrenti, perché non sfugge a nessuno che i sondaggi danno il Movimento 5 Stelle quale primo partito in Italia e candidato a un ruolo di Governo nel prossimo futuro. Se ora si esprimesse in qualche modo contrariamente e debolmente rispetto alla candidatura di Milano, com'è stato fatto ad esempio nel caso della candidatura di Roma alle olimpiadi, questa sarebbe una iattura per l'Italia. Spero che venga confermato nel voto odierno quanto ieri ha indicato, seppure in tutt'altro contesto, il collega Cappelletti, ovvero l'ovvio favore alla candidatura, anche se egli non riteneva utile discuterne in quest'Aula, come pure ha un po' confermato il collega Crimi poco fa. Non è assolutamente così. Il Parlamento, e il Senato in particolare, può e deve fare la sua parte, proprio in vista degli appuntamenti decisivi delle prossime settimane. Entro novembre si decide e l'Italia, che punta tutto su questa prestigiosa sede, in quanto ha presentato la candidatura solo per l'Agenzia europea del farmaco e non per l'altra agenzia (l'Agenzia bancaria europea), non può permettersi dubbi e incertezze. Le candidature concorrenti sono ben 18 - come già detto - e alcune ben posizionate rispetto ai sei criteri oggettivi che sono stati indicati, che ripeto velocemente, per ribadire quanto Milano sia ben posizionata. Il primo è la garanzia che l'Agenzia possa essere istituita *in loco*. Quindi, Milano, avendo messo a disposizione

se lo confrontiamo con quanto esiste in giro per il mondo. Quanto al mercato del lavoro, in Lombardia abbiamo fortunatamente dei tassi di disoccupazione molto più bassi rispetto ad altre realtà italiane e sicuramente tra i più bassi d'Europa.

Voglio aggiungere allora la mia voce a quella dei colleghi che mi hanno preceduto per dire che la Sardegna, che pure è distante da Milano, ritiene che un'Agenzia di questo genere, visto il suo interesse e lo sviluppo che la stessa richiede,

un territorio veramente importante dal punto di vista della ricerca scientifica e farmacologica. Dispiace perché a tutto titolo avremmo avuto la possibilità di competere con altri territori. allora l'invito fatto precedentemente dal collega Crimi: su questa iniziativa cerchiamo di non dividerci. Non oso neanche pensare che ci sia una speculazione da parte di altri territori. Penso che poche volte come questa un'espressione unanime e unitaria di tutto il Senato possa costituire un biglietto da visita positivo per chi ci analizza dall'estero.

la possibilità di far fare un balzo in avanti alla nostra ricerca scientifica per intero, perché l'EMA non agisce come un oggetto estraneo in un territorio. L'Agenzia può essere un'occasione importante

Signora Presidente, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'Agenzia europea del farmaco, che attualmente ha sede a Londra, deve trovare un'altra sede. Noi riteniamo che Milano sia una città più che adeguata per accogliere l'Agenzia per una serie di ragioni: l'area della grande Milano genera un PIL da 153 miliardi di euro e, con l'indotto regionale, 359 miliardi Nell'area operano 3.600 multinazionali. Milano è un polo farmaceutico internazionale: sono oltre 200 le aziende produttrici di medicinali; 64.000 le persone impegnate direttamente nel settore; 30 miliardi il il valore produttivo e 2,7 miliardi l'investimento (dati di Farmindustria). Inoltre, Milano ha già la sede praticamente pronta - il Pirellone che, con qualche adattamento strutturale, è immediatamente operativo - ed è una grande città in grado di accogliere le famiglie dei 700-800 dipendenti, con tutto quel che ne consegue. Inoltre, Milano è una città fortemente infrastrutturata, con 2 aeroporti, 350 voli al giorno, treni, reti informatiche, eccetera. nel suo territorio molte attività complementari di ricerca biomedicale e biotecnologica, con 8 università, 17 istituti scientifico-ospedalieri e 32 centri di ricerca. L'alto livello di ricerca italiana viene riconosciuto come uno dei migliori nelle classifiche mondiali. L'Italia, infatti, si posiziona al settimo posto al mondo per numero di studi prodotti nell'ambito delle biotecnologie. Per tutte le ragioni esposte, riteniamo quindi che Milano sia davvero la sede ideale. Un'ultima cosa che intendo sottolineare è proprio il fatto che la nostra candidatura è già stata perorata lo scorso 25 settembre,

che il Governo e il Parlamento sapranno mettere in atto tutte quelle situazioni di trasparenza nella gestione di un'Agenzia così delicata. Auspichiamo davvero che il Governo sappia mettere in campo tutto il suo peso in ambito europeo per il buon esito del trasferimento dell'Agenzia

È stato un peccato che la mozione presentata il 2 febbraio 2017, proprio dal senatore Mandelli - come è stato ricordato poco fa dal collega che mi ha preceduto

sul trasferimento della sede dell'EMA. Ora siamo verso la volata finale, perché nell'arco di un mese, dopo una prima scrematura tra le città che si sono candidate, si sceglierà tra una rosa di tre. Quindi, entro il

Bucarest, Copenaghen, Dublino, Helsinki, Lille, Porto, Sofia, Stoccolma, Malta, Vienna, Zagabria e Varsavia.

a Bruxelles per spingere Milano nella corsa ad aggiudicarsi EMA, l'Agenzia europea del farmaco. C'è stato un importante evento, organizzato da Confindustria, Farmindustria, Federchimica, la Fondazione Milano per Expo 2015, la Camera di commercio Milano-Monza-Brianza-Lodi e Assolombarda, per presentare alla *business community* europea tutti i punti di forza della candidatura italiana.

il tessuto industriale, di ricerca e di produttività, nonché la logistica e i trasporti, Milano offre di più, e non ne abbiano contro di me i colleghi pugliesi. Spero che non si applichino strani criteri di equilibrio geopolitico: si parlava di un asse Macron-Merkel per dividersi le due Agenzie: quella del farmaco in Francia e quella bancaria Mi auguro che il Governo, forte di tutto questo sostegno e delle ragioni oggettive nel criterio della scelta della sede di un'Agenzia importante come quella del farmaco,

Come è stato ricordato anche nell'ultimo intervento, a seguito del *referendum* di separazione della Gran Bretagna dall'Unione europea nel giugno 2016,

europea). Da subito il Governo precedente e l'allora presidente del Consiglio Renzi hanno assunto l'iniziativa per candidare Milano a sede per l'Agenzia europea per il farmaco, latori in quel caso di un'indicazione corale delle principali istituzioni interessate: oltre al Governo, la Regione Lombardia e il Comune di Milano. Ma voglio ricordare - e la collega Rizzotti ha ragione ragione - anche il mondo della ricerca e dell'imprenditoria milanese e lombarda, che hanno dato un contributo rilevante e di sostegno sostegno all'assunzione di questa iniziativa. Il 13 settembre 2016 il il progetto EMA-Milano è stato inserito nel patto per la Lombardia che l'allora presidente del Consiglio Renzi ha firmato con il presidente della Regione Maroni.

per segnalare l'intensità con cui questa partita importante e delicata, come evidenziato dalla collega De Biasi, è stata seguita è stato istituito un tavolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, presieduta dal professor Moavero Milanesi e composta da tutte le principali istituzioni: il Ministero per gli affari esteri, il MIUR, il MISE, il Ministero della salute, la Regione Lombardia e il Comune di Milano. Intensa è stata quindi l'attività a sostegno e in particolare l'attività diplomatica che è ancora in corso, a partire dall'azione - anch'essa testé ricordata - del Presidente del Consiglio. Ultima iniziativa è l'incontro di lunedì scorso a Bruxelles dove la ministra Lorenzin, insieme al presidente Maroni, al sindaco Sala e al professor Moavero Milanesi hanno presentato la candidatura di Milano. Sabato ci sarà una prima valutazione delle offerte di candidatura. A cavallo del 20 novembre sarà presa la decisione finale da parte di organismi europei che - immagino a margine del Consiglio europeo del 19 e del 20 ottobre tratteranno la questione. Io penso che l'unità istituzionale e politica del Paese sia fondamentale per tentare di raggiungere questo obiettivo.

l'iniziativa italiana in relazione al Consiglio europeo dei giorni successivi. Mi auguro che anche quella sia la sede, al di là delle divergenze politiche, per ribadire l'unitarietà di intenti e rafforzare il mandato del Governo e del Presidente del Consiglio. Come veniva ricordato, l'EMA ha 890 dipendenti, diversi comitati scientifici e opera con migliaia di esperti e ricercatori, sia sul tema del nuovo farmaco che sul tema del monitoraggio della qualità dei farmaci presenti in commercio. I temi della qualità del farmaco e della qualità della salute sono strettamente connessi e sono una delle ragioni importanti per cui è stata avanzata la candidatura di Milano. Potremmo dire che Milano è la città vocata per essere sede, non solo perché corrisponde a tutti criteri individuati per l'assegnazione, ma anche perché si trova in un Paese, l'Italia, che, con la Germania, è il primo produttore di farmaci in Europa e, per di più, nel cuore di un polo di studi, di ricerca e di produzione tra i più qualificati al mondo. Oltre ai numerosi punti di forza contenuti nel *dossier* che il tavolo di coordinamento ha preparato in sede di Presidenza del Consiglio, d'intesa con la Regione Lombardia e con il Comune di Milano,

Questo è un grande punto di forza sulla qualità del sistema Paese. Il secondo - del quale voglio ringraziare in modo particolare il presidente Maroni - è l'aver messo a disposizione un luogo prestigioso come sede della nuova Agenzia. Agenzia. Avere la sede a disposizione è un grande punto di forza, perché solo noi e Barcellona

dato dalla Regione Lombardia e anche dal Comune di Milano una grande azione di sostegno. Ringrazio il Parlamento, nella fattispecie il Senato, per l'azione di sostegno all'iniziativa del Governo e delle diverse istituzioni, che, in realtà, è un'azione di sostegno al Paese nel nome nel nome dell'interesse generale e dell'interesse nazionale. Mi auguro che ciò si concluda con un voto unitario sulle diverse mozioni e venga ribadito, appunto, alla presenza del Presidente del Consiglio mercoledì 18

con la soppressione di «a seguito dell'intuizione e proposta del presidente della Regione Maroni» perché - come ho già spiegato - è un'iniziativa

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1,

e delle città di provincia a mettere una perla strategica in una città metropolitana. È un segnale chiaro e forte del supporto e del contributo che quest'Aula - e il Parlamento intero - vuole dare affinché le negoziazioni per portare l'Agenzia europea del farmaco (EMA) in Italia volgano a buon fine. Colleghi, il voto per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, seppur da un lato rappresenta un processo complicato a causa del quale l'intera comunità dei 27 dovrà subire inevitabili contraccolpi, dall'altro ha reso possibile l'apertura di alcune finestre di opportunità potenzialmente molto interessanti per il nostro Paese, che dobbiamo cogliere. Penso all'EMA, ma anche ad altre possibili Agenzie e opportunità quali - ad esempio - un'Autorità europea per la tutela degli animali o dei monumenti storici e per la strategia per la prevenzione sismica

Poter ospitare queste autorità sul nostro territorio, nelle nostre città, non solo costituisce un motivo di vanto istituzionale, ma si traduce anche nella creazione di un indotto dal punto di vista occupazionale, della ricerca, dello sviluppo e ci aiuta a rendere maggiormente attrattivo - dal punto di vista economico - il Paese intero. Solo per fare un esempio, l'EMA organizza in media 500 incontri internazionali all'anno che mettono in movimento 500.000 persone. Non è un caso che molte società farmaceutiche avessero, negli anni scorsi, stabilito sedi a Londra per essere vicine a EMA. probabile che decideranno di spostare le loro filiali nella città che sarà scelta per ospitarla in futuro, creando un'ulteriore crescita. Per questo è oggi più che mai importante fare squadra. Lo dico pensando a una sinergia positiva tra istituzioni, settore produttivo, università e ricerca; lo dico, colleghi, anche pensando con un po' di amarezza ai recenti casi di altre città, tra cui Roma, la cui amministrazione non ha avuto il piglio e la lungimiranza per comprendere questa opportunità, trasformandola nell'ennesima occasione persa. Tornando a Milano, oggi è arrivato il momento di mostrare sul tavolo della trattativa con la Commissione e il Consiglio europeo che il prossimo novembre dovranno scegliere il candidato vincitore che non si tratta di Milano, ma del nostro sistema Paese. Non possiamo puntare soltanto sui dati, seppur solidi e in crescita, del settore farmaceutico lombardo; sono molte di più è molto più rilevanti le ragioni per sostenere la candidatura di Milano come prossima sede dell'EMA. Prima di tutto abbiamo un motivo logistico: un'Autorità che ha il compito di autorizzare nuovi medicinali in tutta Europa non può fermare la sua attività nemmeno per un giorno; se ciò avvenisse ne pagherebbero le conseguenze dirette i cittadini e i pazienti. Ecco perché è assolutamente necessario che la nuova sede sia pienamente operativa in tempi brevissimi e che sia anche inserita in un tessuto socioeconomico e scientifico adeguato, che possa supportare il cambiamento, garantendo la giusta continuità. A Milano ci sono gli uffici già pronti e infrastrutturati messi a disposizione dalla Regione Lombardia, cioè il grattacielo Pirelli, disegnato più di sessant'anni fa da Giò Ponti, Pier Luigi Nervi e altre *archistar*. Per il trasloco è sufficiente staccare le spine dei *computer* nell'edificio dei Docks di Londra e riattaccare le prese nel grattacielo di via Fabio Filzi. Inoltre, si sta già lavorando per l'apertura di uno sportello per assistere il trasloco e gli addetti EMA in tutte le loro necessità. Oltre all'infrastruttura fisica e alla disponibilità di spazi, contano i tempi e le distanze dei collegamenti con treni ad alta velocità e aeroporti, la capacità ricettiva per dipendenti, visitatori, partecipanti ai grandi eventi internazionali e Milano, soprattutto a seguito di Expo, può dirsi pronta. ho anche un po' di amarezza, perché penso ad esempio alle Marche, che potrebbero essere centro della macroregione adriaticoionica e che però non sono collegate così bene, anzi, dal punto dal punto di vista infrastrutturale sono un po' il fanalino di coda di questo Paese. Investire nelle infrastrutture è importante; spesso si fanno delle battaglie contro che sono ideologiche, ma i collegamenti aiutano anche in una prospettiva di sviluppo verde, perché ridurre i percorsi e i tempi significa anche impattare meno dal punto di vista delle emissioni ambientali. oltre all'infrastruttura fisica e alla disponibilità di spazi, contano i tempi e le distanze dei collegamenti con treni ad alta velocità e aeroporti. Questo è importante, perché Milano è pronta. non si possono tralasciare altri elementi non misurabili con il sistema metrico decimale, ma fondamentali. Penso agli elementi espressi dall'ambiente culturale e sociale circostante: per esempio, l'industria italiana del biomedicale, dei principi attivi farmaceutici e delle biotecnologie. Penso all'università di Bologna che sta studiando dei brevetti che sarebbe importantissimo finanziare, perché questo la farebbe tornare ad essere città dell'eccellenza, dei brevetti

Questa rete potrebbe costituire un polo scientifico di cooperazione per la ricerca unico in ambito continentale, abbracciando settori importanti e correlati tra loro, quali la scienza della vita, dell'alimentazione e della nutrizione. Insomma, a Milano piace vincere facile in questo caso, perché le condizioni ci sono tutte e potrebbe diventare quel cuore pulsante che ci farebbe piccoli sì, ma grandi in Europa. Colleghi, questi sono i motivi per cui vale la pena sostenere la candidatura di Milano e farlo con convinzione. Occorre farlo non solo per Milano, ma per l'Italia.

Non può occuparsi di argomenti così importanti a livello strategico chi non lo ha fatto e spero che non occorra il bollino blu della Casaleggio Associati per essere in regola in questo caso. Spero che i parametri di trasparenza siano altri e valgano per il Paese e per tutti. Ci sono battaglie politicodiplomatiche che misurano più di altre lo *standing* internazionale di un Paese e quella per aggiudicarsi la sede dell'EMA è una di queste.

Sappiamo però che c'è il problema dei concorrenti e delle altre città che si sono fatte avanti ed è qua che diventa essenziale il peso del Governo.

effettivamente tutte le motivazioni per cui si vuole Milano e non Bratislava. La cosa che ci sta preoccupando è che purtroppo, invece, si

Mi auguro veramente che da qui a quando decideranno, a novembre, si riescano a trovare la forza e la determinazione che il Governo deve avere per portare la sede dell'EMA a Milano.

al principio di favorire la presenza di fronte alla stazione centrale di Milano di questa importante sede, ma ritengo che non sia dirimente il fatto che

pali e paletti, bisogna farla venire punto e basta. Non è per una sede che si può parlare di cementificazioni. La sede c'è già

che riguardano anche la sede degli enti di regolazione del farmaco, rispetto ai quali l'Italia ha buona parte delle carte in regola per potersi presentare con una forte candidatura.

che spesso non abbiamo brillantemente presenti nella nostra realtà, nella gestione delle politiche del farmaco e nel governo dell'industria farmaceutica, che certamente, in qualche caso, a livello internazionale non ci fanno apparire al primo posto nella compagine dei Paesi europei. Questa, però, è anche una grande occasione per imparare ad assumere trasparenti e di rispetto del controllo dei conflitti d'interesse che forse non abbiamo sempre tenuto in maniera sufficientemente chiara. Mi auguro davvero, quindi, che se questa candidatura andrà a buon fine, sia anche utile per adottare uno stile,

Credo che esse siano finalizzate a sostenere le ragioni del tricolore e indubbiamente tali ragioni devono portarci ad un atto di responsabilità, abbandonando la logica del campanile e seguendo una strada maestra, che ci porti a selezionare ed a sostenere in Italia la sede oggettivamente più idonea in termini di requisiti Ritengo che le candidature che sono state presentate - come auspicio, perlomeno - da varie sedi nazionali siano tutte rispettabili

alla valutazione del decisore sovranazionale con una proposta credibile, la migliore possibile,

Credo che il valore simbolico di questo voto, che sono convinto consegnerà una valutazione ed una visione unanime, dia forza all'auspicio all'auspicio di fare in modo che le valutazioni che si faranno per la scelta vedano prevalere le condizioni logistiche e tecniche rispetto a quelle politiche. Per carità, mi rendo conto che la diplomazia internazionale è al lavoro perché anche le sfumature politiche non siano estranee alla scelta, ma credo che sia necessario

in regola e le condizioni per rappresentare il tricolore nazionale in una versante nel quale l'Italia è un'eccellenza. Non dimentichiamo che l'AIFA è l'agenzia regolatoria del farmaco nazionale più qualificata, più accreditata e più considerata a livello mondiale e non a caso il presidente dell'EMA è un italiano, il professor Guido Rasi, sulla cui credibilità, sul cui talento e sulla cui competenza scientifica credo ci siano valutazioni unanimemente positive.

assolutamente adeguata alla sfida che va affrontata con la sede dell'EMA nel capoluogo lombardo. Vi è inoltre la presenza di infrastrutture scolastiche e di assistenza sanitaria, riguardo alle quali Milano certamente dimostra di essere un'eccellenza a livello europeo. Ma non ci sono soltanto le valutazioni di tipo logistico e le valutazioni relative alla capacità di assorbire con grande efficienza il traffico internazionale dei trasporti convergente su Milano e che parte da Milano per gli altri Paesi dell'Unione. Il tema merita di essere esteso, con una valutazione, anche al fatto che l'Italia può vantare la sua posizione di secondo Paese nell'ambito della produzione di farmaci in Europa, dopo la Germania, il tasso di esportazione di farmaci dall'Italia non ha rivali, perché si tratta di una percentuale senza pari, con un riconoscimento assoluto che ci viene a livello internazionale per la qualità e le competenze di tutti gli addetti. evidenziato anche quanto, nell'area biotecnologica, l'Italia abbia punte di eccellenza a livello mondiale, che probabilmente noi

accrescimento culturale e di una spinta energica che l'EMA può determinare in Italia, non soltanto nell'ambito del territorio lombardo, ma in tutto il Paese. il Paese. Concludo dicendo che l'impegno assunto dal Governo su questo versante è stato efficace e tempestivo, perché l'aver stanziato 54 milioni di euro per la realizzazione della sede dell'EMA a Milano è un segno evidente di attenzione e di energica affermazione di una volontà con cui ci si presenta nel panorama europeo con le carte in regola e con una volontà granitica e unanime del Paese, senza se e senza ma. La raccomandazione con cui concludo è che gli effetti indubbi di beneficio le ricadute sotto il profilo economico, culturale e scientifico rivenienti dall'EMA in Italia, a Milano, devono poter rappresentare un beneficio senz'altro per l'area del distretto milanese e lombardo, ma anche per tutto il Paese, tentando di coinvolgere, attraverso un virtuosismo operativo, quelle parti del Mezzogiorno d'Italia che sono esse stesse punti di eccellenza nell'ambito di questo comparto. Alla luce di queste osservazioni e di queste motivazioni e apprezzando molto lo sforzo che è stato fatto tramite le mozioni e la sintesi che in esse viene fatta di tutta questa tematica, con una nota di particolare apprezzamento per il lavoro svolto dal collega senatore Mandelli, annunzio il voto convintamente favorevole su tutte le mozioni da parte dei senatori del Gruppo

cercherò di essere breve. Mi fa molto piacere che si stia andando, come mi sembra di capire, verso un voto unanime per la candidatura di Milano; non lo davo per scontato e questo mi fa piacere. Vorrei fare solo qualche appunto su quanto ho sentito. In particolare, ha segnalato un problema con cui concordo, sull'attenzione al tema della possibile presenza dell'attività di portatori di interesse, sia pubblici che privati, nel rapporto con l'Agenzia: direi che

il registro delle *lobby*, intanto che esso diventi obbligatorio, essendo attualmente applicato solo al Parlamento europeo e alla Commissione europea; si chiede che venga esteso anche al Consiglio europeo e, a questo punto, aggiungerei anche alle Agenzie.

è già ben definito e ci potranno essere più scrutini; al primo scrutinio, ogni Paese ha sei voti a disposizione, da assegnare a tre città candidate,

In questo momento, con le mozioni in esame, diamo forza ad un'iniziativa che il Governo, in maniera meritoria, sta portando avanti,

E questo sicuramente sarebbe un grandissimo onore per l'Italia. Quindi, non ci dovrebbero e non ci possono essere divisioni di sorta. Possono esserci sensibilità diverse? Certamente sì, ma dobbiamo raggiungere l'obiettivo tutti quanti insieme. Bene hanno fatto i parlamentari della Lombardia a riunirsi e a fare corpo comune per vincere questa battaglia; bene hanno fatto i parlamentari europei italiani a fare altrettanto. Bene hanno fatto la Regione, il Comune e la Provincia della Lombardia e bene facciamo noi a a stringerci intorno al Governo in questa grande battaglia. Colleghi, avere l'EMA in Italia non è cosa di poco conto, lo hanno già detto i colleghi e lo voglio ribadire. L'EMA in Italia significa un potenziamento straordinario di tutta quella filiera industriale del farmaco e della ricerca rispetto alla quale noi siamo principi in Europa e nel mondo.

in casa nostra significa non soltanto avere ricercatori, grandi potenze scientifiche e tutto ciò che ne consegue, ma anche avere un substrato culturale enorme che dobbiamo accogliere a piene mani. Perdere questa opportunità sarebbe come perdere un'occasione strategica, e sappiate, colleghi, che se la perdiamo soltanto perché qualcuno pensa di poter lucrare sulla sconfitta dell'Italia

mozioni oggi al nostro esame siano importanti, non banali e non ovvie. Sono importanti perché dicono che il Parlamento, e in particolare il Senato della Repubblica, è insieme al Governo, agli enti e a tutti coloro che su questa battaglia stanno mettendo il loro impegno. Ci siamo anche noi, vogliamo esserci da qui fino alla soluzione del problema. problema. Vogliamo festeggiare insieme alla Lombardia un grandissimo risultato che, non soltanto per la Lombardia, ma per i nostri ricercatori, per la nostra Italia, per tutti quanti noi sarebbe motivo di grande vanto. Voteremo assolutamente in modo conforme a tutte le indicazioni che anche il Governo oggi ci ha dato relativamente alle mozioni presentate. *(Applausi Signor Presidente, anche Sinistra Italiana voterà a favore

Lombardia; noi, ad esempio, avevamo proposto la possibilità di utilizzare il sito EXPO a Milano, ma l'importante è comunque evitare la proliferazione di infrastrutture anche perché l'area milanese è ampiamente dotata, com'è stato detto in tantissimi interventi e dai parlamentari lombardi, di ricchezze particolari anche da questo punto di vista. Sicuramente noi appoggiamo e sosteniamo il lavoro che stanno facendo il Governo, le istituzioni

ma non del tutto irrilevante considerazione. Ci auguriamo che il trasferimento della sede dell'Agenzia da Londra a Milano possa essere anche l'occasione per rivedere il ruolo e le modalità operative perché nei suoi anni di attività sono stati tanti i rilievi fatti sulla subalternità agli interessi delle industrie farmaceutiche e soprattutto sulla scarsa trasparenza delle decisioni, proprio per la stretta collaborazione con le industrie produttrici e l'omissione di informazioni utili. Noi pensiamo che, proprio perché si tratta di un'Agenzia che protegge e promuove la salute pubblica attraverso la valutazione e la supervisione dei farmaci che vengono immessi in commercio, i temi della trasparenza dei dati, della conoscenza e soprattutto della terzietà, per evitare conflitti di interesse, debbano essere uno

contribuire a cambiare anche le procedure a tutela della salute pubblica.

Apprezziamo anche la volontà del Governo di accogliere l'ordine del giorno che abbiamo presentato, che ha lo scopo di fare demagogia, come qualcuno ha detto, ma semplicemente di prendere atto di una situazione di fatto e che la Regione Lombardia ha dato la disponibilità di un immobile,

Tra i requisiti è previsto l'accesso al mondo del lavoro per i familiari dei dipendenti e dei tecnici che lavoreranno nell'ambito dell'Agenzia.

questo intervento significa che c'è la possibilità, da parte del Governo, di intervenire

Per il resto ci auguriamo che la trasparenza sia l'elemento chiave in tutte le operazioni che da qui in avanti condurranno alla decisione

e non solo annunci via Twitter, Facebook o comunicati stampa. Ci piacerebbe che siano messi in atto da parte del Governo

sull'EMA, va di pari passo con l'iniziativa che qualche giorno fa le imprese hanno voluto portare a sostegno di questa candidatura. un momento importante proprio a Bruxelles, quando Confindustria, Farmindustria, Federchimica, Fondazione Milano per Expo 2015, camera di commercio di Milano, Monza e Brianza, Assolombarda hanno voluto dare il significativo impulso del mondo del fare, dell'impresa, delle associazioni, che chiedono chiedono che questo voto sia anche interprete della loro volontà di portare l'Agenzia del farmaco in Italia. Credo che con

nelle migliori condizioni per accogliere questa Agenzia così importante. Quindi, questa unità politica alla vigilia di tale sfida, con diciotto città che hanno avanzato una candidatura (tutte autorevoli, anche se personalmente le ritengo inferiori

per tranquillizzarlo), ciò che è importante è che smettere di lavorare in Inghilterra vorrà dire dopo pochi giorni poter lavorare a Milano. Questo è davvero il punto di forza nella continuità dell'operatività che noi possiamo vantare rispetto a tutte le altre candidature.

Continuità operativa, eccellenza, sistema lombardo che funziona e sistema Paese che vuole questa opportunità: è per questo che è importante portare EMA a anche lo sforzo che stiamo facendo per far diventare centrale il nostro Paese nel mondo della ricerca: sto pensando a Human Technopole, che potrà essere un'importante sinergia per valorizzare il lavoro che spero veramente possa essere svolto a Milano.

dall'innovazione. Dobbiamo fare le cose perbene - questo è un altro ragionamento - però dobbiamo accettare anche il rischio di andare avanti, perché ogni cosa nuova può portare dei problemi, ma bisogna vedere come vengono È per questo che, nonostante il contenuto della loro mozione, noi voteremo favorevolmente: perché la sfida vera del Paese non è non fare le cose, ma farle perbene, cercando di fare in modo che tutto sia fatto secondo criteri corretti, nella piena trasparenza e nella piena volontà

considerazioni già risuonate in Aula nella presentazione delle mozioni, nel dibattito successivo e ancora nelle dichiarazioni di voto.

È un atto importante che, certamente, si inserisce in modo funzionale e politicamente valido in un processo, che hanno già ricordato i presentatori delle mozioni ma che ha puntualizzato, molto bene e rigorosamente, il sottosegretario Pizzetti. Il nostro Paese è impegnato, dal giorno dopo la Brexit, a sostenere la candidatura di Milano come sede dell'EMA.

Il farmaco oggi è un elemento in fortissimo cambiamento. Ormai i nuovi farmaci sono delle vere e proprie biotecnologie. Determinano e stressano soprattutto i sistemi nazionali come il nostro, basato sulla solidarietà

allora, c'è bisogno di una politica di *governance* del farmaco, per quello che oggi è diventato il farmaco, all'altezza dei tempi e di questa sfida.

terziaria, del suo ambito di ricerca, possa essere, e sia, la sede più opportuna. Noi abbiamo detto, giustamente, che l'EMA a Milano è una *chance*, certamente per Milano, ed una grandissima *chance* per l'Italia. Io vorrei aggiungere che l'EMA a Milano è una *chance* per l'Europa e per le sue agenzie internazionali. Per

Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione. Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordine del giorno G1

Il relatore, senatore Russo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi non ripeterò quanto detto in questa sede il 18 maggio, quando ho avuto occasione di presentare la legge. Intervengo solo per depositare alcuni emendamenti del relatore,

ci sentiamo tutti in dovere di provare a portare a casa perché siamo l'ultimo Paese in Europa che ancora non ha normato sul tema

strettamente procedurali e solo un paio sono contenutistici. Abbiamo voluto raccogliere quanto emerso in discussione generale già nella prima fase di presentazione del provvedimento in Aula. L'obiettivo è giungere tutti a condividere

stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per uso terapeutico». Ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, la discussione su tale richiesta

Presidente, so che lei è molto attento alle questioni delle telecomunicazioni e la prego di prestare attenzione perché potrebbe aiutare a sensibilizzare ulteriormente il Governo. In questi giorni si sono moltiplicati i blocchi e i picchetti da parte dei sindacati Si Cobas e Sol sigle minoritarie all'interno dei 9.000 lavoratori, diretti e indiretti, della SDA, che stanno producendo una drammatica una drammatica riduzione dell'operatività dell'azienda. Sono già state messe in atto dall'azienda procedure di cassa integrazione

La Polizia, intervenuta casualmente all'inizio dei blocchi, ha fermato un manifestante che stava procedendo al picchettaggio dei cancelli dell'azienda in possesso di un'ascia. possesso di un'ascia. Visto che l'azienda è di proprietà totale di Poste Italiane, e non mi risulta che allo stato attuale Poste Italiane abbia chiesto al Ministero degli interni un intervento deciso per garantire, sì, il diritto di sciopero, ma anche per impedire che questo diritto pregiudichi l'operatività dell'azienda ed il lavoro di 9.000 persone in Italia, prima che accada qualcosa di drammatico davanti a questi stabilimenti, mi aspetto un intervento deciso - e la prego, signor Presidente, di farsi latore di questa richiesta presso il Governo - da parte dei prefetti delle aree interessate, che mi pare stiano aumentando e non diminuendo. Non è accettabile, di sigle minoritarie, a cui nessuno nega il diritto di manifestare, anche se non è chiaro quali siano le ragioni dello sciopero, perché francamente ho avuto modo di parlare con i sindacati confederali e nessuno capisce qual è

sono stati arrestati mentre prendevano una tangente da un'impresa per far terminare lo sciopero. Chiedo quindi un intervento immediato da parte del Ministero dell'interno. alcuni mesi fa abbiamo presentato la richiesta al Ministero dell'interno di valutare la possibilità di accedere al mercato di Vittoria, ai sensi della normativa antimafia. di qualche giorno fa la notizia che nell'operazione «Exit poll» la Guardia di Finanza ha eseguito delle ordinanze di custodia sull'ex sindaco del Partito Democratico e sul consigliere suo fratello, Giuseppe Nicosia e Fabio Nicosia, i quali, in contatto con esponenti della criminalità organizzata, sarebbero incorsi nel reato di scambio politico-mafioso.

Tutto questo avviene in una situazione di imbarazzo per il Partito Democratico, in una situazione di imbarazzo per il centrodestra, perché il sindaco è uno dei sostenitori del candidato Presidente del centrodestra in Sicilia, ed avviene nel silenzio del Movimento 5 Stelle vittoriese (tra l'altro non siamo abituati al silenzio del Movimento 5 Stelle e la cosa ci appare un po' curiosa).

per la situazione di crisi dell'agricoltura, indotta anche dai rapporti con la grande distribuzione organizzata, sia per una serie di attentati di chiara matrice mafiosa, sia per una situazione strana per la quale gli immobili posti a garanzia ipotecaria dei prestiti richiesti dagli agricoltori vittoriesi vengono regolarmente venduti a a prezzi vili, creando condizioni per le quali queste persone arrivano alla rovina assoluta, perdendo i propri beni immobili e rimanendo ancora debitori.